Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, l'articolo 36 della legge di contabilità e di finanza pubblica affida al Rendiconto generale dello Stato il compito di rendicontare al Parlamento, nella forma della legge, l'avvenuto rispetto di quanto autorizzato con la legge di bilancio. L'approvazione del Rendiconto generale dello Stato rappresenta, pertanto, l'atto conclusivo del processo di bilancio, attraverso cui le Camere prendono atto delle risultanze contabili scaturenti dalla gestione avvenuta nell'esercizio precedente. Sul piano procedurale e tecnico contabile, la stessa proposta di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2017, il cui esame verrà avviato nei prossimi giorni in prima lettura alla Camera, assumerà quale base di riferimento le risultanze definitive contenute nel Rendiconto, le quali sono state altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2016, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento. Il Rendiconto, alla stregua del bilancio, è articolato in missioni e programmi ed è composto dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite previste dal bilancio dello Stato dell'anno precedente, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nelle attività e nelle passività che costituiscono il patrimonio dello Stato, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. Al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati. Il Rendiconto medesimo è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. In relazione al contenuto del provvedimento, si evidenzia che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 e sono riferiti rispettivamente alle entrate, che troverete nel dettaglio nella relazione. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2015, un disavanzo di 245.428,1 milioni di euro. L'articolo 5 reca l'approvazione dell'allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste», nonché l'approvazione dell'allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2015, da cui risultano attività per un totale di 962,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.721 miliardi di euro. Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome. Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome, secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti. Nel merito, passando ai dati complessivi del bilancio dello Stato, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2015 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive. In particolare, il saldo netto da finanziare presenta nel 2015 un valore pari a meno 41.545 milioni di euro, con un miglioramento di 11.294 milioni rispetto al saldo registrato nel 2014, dovuto al buon andamento delle entrate finali. Analizzando l'andamento delle entrate e delle spese correnti, si evidenzia, invece, l'ulteriore netta flessione registrata dal risparmio pubblico che, dopo essere sceso nel 2014 a 18,4 miliardi di euro rispetto ai 39,7 miliardi del 2013, si attesta nel 2015 ad un valore negativo di 9 miliardi di euro, dovuto ad un forte incremento delle spese correnti rispetto al 2014 (di oltre 43 miliardi), riconducibile ad una impostazione meno rigida di politica fiscale nel corso del 2015, solo in parte compensato dall'incremento delle entrate correnti (+16,1 miliardi). Anche in questo caso il risultato è comunque migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più negativi (oltre i 33 miliardi Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (ossia la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2015 sulla cifra di 257,1 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, 2015, che risultava fissato in meno 70.884 milioni per il saldo netto da finanziare e in meno 323.000 milioni per il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse. Il miglioramento del saldo netto da finanziare sopra evidenziato discende da una gestione di competenza che mostra un'evoluzione positiva dell'andamento degli accertamenti di entrate finali rispetto al 2014, per la maggior parte ascrivibile alle maggiori entrate tributarie accertate, i cui effetti positivi risultano in parte compensati da un aumento moderato degli impegni di spesa. L'andamento crescente delle entrate finali accertate sarebbe riconducibile, oltre che al miglioramento del ciclo, all'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - riguardante la semplificazione fiscale e l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata che ha modificato i meccanismi di compensazione e restituzione delle imposte tributarie. Dal lato della spesa, un orientamento meno restrittivo della politica di bilancio ha determinato un incremento complessivo degli impegni finali, in particolare della spesa corrente (più 43 miliardi di euro rispetto al 2014), cui ha fatto peraltro riscontro la riduzione della spesa in conto capitale (meno 35 miliardi

Tale andamento rispetto all'esercizio 2014 trae origine dalla dinamica dell'accensione di prestiti, che ha registrato una contrazione di oltre 30 miliardi di euro (meno 10,4 gli impegni complessivi di spesa ammontano a 826.631 milioni di euro. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta un aumento complessivo degli impegni di spesa di 16 miliardi di euro (più 2 Nel complesso, il peso della spesa complessiva in rapporto al PIL è passato dal 50,2 per cento del 2014

L'aumento delle entrate finali trova giustificazione nella crescita del PIL che ha determinato principalmente un aumento del primo titolo delle entrate. Rispetto al 2014, infatti, si registrano un aumento delle entrate tributarie (che si attestano intorno ai 477,2 miliardi di euro) e una flessione delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 83,6 miliardi di euro. Le entrate relative al Titolo III «Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti» registrano un aumento di 3,2 miliardi di euro rispetto al 2014. L'analisi in dettaglio delle singole componenti gestionali che hanno concorso alla dinamica di competenza mostra, dal lato delle entrate, che le entrate tributarie si attestano sulla cifra di 477.178 milioni di euro

Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i recuperi, rimborsi e contributi (-1,2 miliardi rispetto al 2014, pari al -2,6 per cento) e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (-659 milioni rispetto al 2013, pari al -11 In miglioramento per circa 1,4 miliardi di euro sono invece i proventi dei servizi pubblici minori (+5,6 per cento). Notevole, infine, è l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 5,5 miliardi di euro del 2014 agli 8,7 miliardi del 2015, superando il livello dei 7,9 miliardi registrato nel 2012. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni, i quali hanno più che raddoppiato gli introiti. Venendo poi alle spese finali, la gestione di competenza 2015 ha dato luogo - come detto - a impegni di spesa per complessivi 611.111 milioni di euro, in aumento di 8.086 milioni rispetto all'esercizio precedente. In merito, si osserva come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 569.801 milioni di euro (in aumento dell'8,3 per cento rispetto al 2014), mentre quella in conto capitale è scesa a 41.310 41.310 milioni di euro (in diminuzione del 46,2 per cento rispetto al 2014). Con riferimento alla dinamica delle spese correnti, complessivamente aumentate dell'8,3 per cento, confrontando i dati con quelli dell'esercizio 2014, la categoria che registra maggiori aumenti è quella relativa alle poste

Gli impegni per redditi da lavoro dipendente, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni, ammontano a 86.966 milioni di euro, in sostanziale stabilità rispetto La spesa corrente del 2015 si caratterizza poi per una sostanziale stabilità nei consumi intermedi, che passano dai 12,3 miliardi del 2014 ai 12,9 miliardi del 2015 e per un calo degli oneri per interessi passivi, pari a 74,5 miliardi di euro (rispetto a 81,1 miliardi nel 2014 e ancora superiori negli anni precedenti). Sostanzialmente stabili risultano le altre voci. Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano una forte diminuzione, da 76.830 milioni del 2014 a 41.310 milioni 41.310 milioni del 2015 (circa 35 miliardi in meno). La contrazione della spesa in conto capitale rispetto al 2014 è da mettere in relazione al fatto che tale titolo di spesa aveva registrato un notevole incremento nel biennio 2013-2014, per la forte immissione di liquidità nel sistema economico determinata dai decreti-legge nn. 35 e 102 del 2013, con i quali è stata operata una consistente azione di sostegno all'economia e alla domanda interna, volta a favorire lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori. Passando poi alla gestione dei residui, in base ai dati forniti nella relazione al Rendiconto, al 1° gennaio 2015 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti, per un valore complessivo di 209.126 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 113.254 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti,

Nel corso dell'esercizio 2015, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2015 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui. Infatti, rispetto allo *stock* di 209.126 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2015 ne sono stati accertati 150.680 milioni, di cui solo 37.773 milioni incassati e 112.907 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 95.352 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2015, pari a 208.260 milioni. Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 113.254 milioni di residui indicati al 1° gennaio 2015, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 99.304

Non considerando i residui relativi al Titolo III, «Rimborso delle passività finanziarie», pari a 3.340 milioni di euro, i residui passivi delle spese finali ammontano quindi a 109.691 milioni

Nel Rendiconto sono poi esposte e illustrate le risultanze relativa alla gestione di cassa. Va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2014. Il disegno di legge di Rendiconto espone infine il conto generale del patrimonio che - si rammenta - costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2015 emerge una eccedenza passiva di 1.758,4 miliardi

Nel complesso, le risultanze del Rendiconto evidenziano i risultati della strategia di programmazione economica di natura pluriennale che il Governo si è dato contestualmente al suo insediamento nel 2014. I principali obiettivi di questa strategia sono il rilancio della crescita e dell'occupazione, attraverso un'azione di riforma strutturale e di stimolo agli investimenti, sia pubblici che privati, un'impostazione della politica di bilancio favorevole alla crescita, in un quadro di consolidamento delle finanze pubbliche, così da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, la riduzione del carico fiscale e la maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni, così come è obiettivo del Governo il miglioramento della capacità competitiva del nostro Paese. Salto qualche particolare e mi avvio Proprio su questi aspetti il Governo italiano ha avviato da tempo un confronto continuo, serrato e costruttivo con la Commissione europea, finalizzato a consolidare a livello europeo l'azione di sostegno alla creazione di occupazione attraverso un'incentivazione alle politiche di investimenti e riforme che cambino in modo strutturale le potenzialità del nostro Paese e una gestione responsabile delle finanze pubbliche. Questi sono punti a cui non abbiamo mai rinunciato, con l'obiettivo appunto di far ritornare a crescere l'economia a ritmi più serrati e al contempo a rispettare il percorso di riduzione del debito pubblico italiano. Più in generale, comunque, il controllo esercitato dal Governo sui conti pubblici e la serietà oggettiva riconosciuta rispetto al percorso di riforme ci permetteranno di inserire all'interno della prossima legge di bilancio sicuramente misure in favore della crescita e ulteriori interventi a tutela delle categorie più colpite colpite dalla crisi, come lo sblocco dei contratti, i tagli ai contributi per le partite IVA non iscritte agli ordini, il *bonus* per la formazione di insegnanti, i contributi alle pensioni minime, la flessibilità, l'incremento delle risorse per il contrasto alla povertà. Si continua naturalmente e coerentemente con l'azione del Governo rispetto all'assunto che questo nostro Paese ha bisogno di crescita e di investimenti e credo che questo sarà il dibattito che caratterizzerà la prossima manovra di bilancio.

ed è corredato di tabelle e allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa. Per quanto riguarda le previsioni assestate in termini di competenza per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2016, il disegno di legge di assestamento evidenzia un miglioramento del ricorso al mercato e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del risparmio pubblico e dell'avanzo primario. Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a quasi 1,1 miliardi, derivanti da un peggioramento di un miliardo per atti amministrativi e da un miglioramento di 243 milioni associato alle proposte dell'assestamento stesso e ascrivibile a una importante riduzione della spesa per interessi compensata da una riduzione delle entrate finali (in particolare tributarie) e da un aumento delle spese primarie. Ne risulta che tale saldo, nelle previsioni assestate, si attesta su di un valore di -35 miliardi e 355 milioni e, dunque, poco al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in -35 miliardi e 400 milioni di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, è dovuto a un aumento delle spese finali per complessivi 380 milioni di euro e a una riduzione delle entrate finali di circa 715 milioni. Più in particolare, con riferimento al saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, si fa presente che l'incremento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio è dovuto a variazioni positive per atto amministrativo, ascrivibili sia alle spese primarie che alle spese in conto capitale. Per contro, la proposta di assestamento prevede una riduzione delle spese finali (quasi -2,1 -2,1 miliardi), su cui influisce la riduzione della spesa per interessi (poco meno di -4,7 miliardi), che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli pubblici e la riduzione degli interessi passivi sui conti sui conti correnti di Tesoreria (per 1 miliardo). La riduzione delle entrate è dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (poco più di -1,8 miliardi) e riguarda esclusivamente le entrate tributarie (3,5 miliardi circa), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2016 contenute nel DEF dell'aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi di quest'anno. In merito alle entrate finali, il provvedimento al nostro esame propone una riduzione per 1 miliardo e 838 milioni come risultato di una contrazione delle entrate tributarie per 3 miliardi e 510 milioni, di cui 2 miliardi e 129 milioni riferite alle imposte dirette e 1 miliardo e 381 milioni per quelle indirette di un incremento di quelle extratributarie per 1 miliardo e 670 milioni, che deriva principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia, ai dividendi dovuti dalle società partecipate, nonché ai proventi dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche, a seguito della gara di assegnazione stabilita dalla legge di stabilità per il 2015. Si fa presente che gli andamenti del gettito ipotizzati tengono conto dei dati rivenienti dall'autoliquidazione delle imposte nell'anno in corso. Con riferimento, invece, al risparmio pubblico le previsioni assestate sono peggiorative, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 173 milioni. I dati relativi al ricorso al mercato evidenziano nel complesso un impatto positivo sul saldo pari a circa un miliardo e 619 milioni, passando da circa - 256,9 miliardi di euro a circa - 255,3 miliardi. In merito alle spese finali, le variazioni proposte comportano una riduzione di 2 miliardi e 81 milioni che riguardano principalmente - come detto - gli interessi. Con riferimento invece alle previsioni assestate in termini di cassa per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, si osserva, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi. L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 8,9 miliardi, quello del risparmio pubblico di poco più di 2 miliardi, mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 9,3 miliardi, raggiungendo l'importo di oltre 330 miliardi; l'avanzo primario, infine, partendo dal valore negativo di quasi 14 miliardi, giunge ad un importo ugualmente negativo di poco meno di 27,4 miliardi, con un peggioramento percentuale superiore al 96 L'andamento divergente dei saldi di cassa di parte corrente rispetto a quelli di competenza viene attribuito a una pluralità di fattori. In particolare, con riferimento alle spese correnti, alle ulteriori risorse da destinare alle Regioni per il pagamento di residui passivi relativi alla compartecipazione IVA, alle maggiori dotazioni sui capitoli di trasferimenti alle imprese per i lavoratori portuali e per le Ferrovie dello Stato, ai maggiori trasferimenti all'INPS per 774 milioni. In relazione alle spese in conto capitale, invece, esso è associato a contributi agli investimenti ai Comuni per un miliardo e 324 milioni, di cui 737 milioni per l'Aquila e i Comuni del cratere danneggiati dal sisma, 560 milioni in favore del Comune di Roma e altresì ai maggiori contributi agli investimenti alle imprese per 1 miliardo e 183 milioni, di cui 1.000 milioni per le Ferrovie dello Stato. Rilevano, infine, acquisizioni di attività finanziarie per 759 milioni. Passando ai residui passivi, al 31 dicembre 2015, essi ammontano a 109,7 miliardi dei quali 63 di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, mentre 46,7 miliardi provengono dagli esercizi precedenti. La riduzione di circa 3 miliardi dei residui passivi finali, rispetto alla consistenza dell'anno precedente, è riferibile esclusivamente alla sensibile contrazione dei residui di conto capitale (-10,2 miliardi), parzialmente compensata dall'incremento di quelli di parte corrente (7,1 miliardi). I residui di nuova formazione rappresentano circa il 57 per cento del totale, si attestano a poco più di 63 miliardi di euro e registrano una riduzione rispetto all'anno precedente con riferimento sia alla parte corrente che al conto capitale (in misura, rispettivamente, di quasi 1,2 miliardi e di oltre 12 miliardi rispetto ai dati del 2014). Le voci più rilevanti nella formazione dei residui di parte corrente si riferiscono ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai consumi intermedi e ai trasferimenti correnti a imprese. i residui in conto capitale i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, quelli agli investimenti alle imprese, gli investimenti fissi lordi, altri trasferimenti in conto capitale, le acquisizioni di attività finanziarie. Prendendo infine in esame le singole disposizioni del disegno di legge di assestamento, esse intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l'esercizio 2016. In particolare, l'articolo 2 modifica la legge di bilancio disponendo che, al comma 3 dell'articolo 2, la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici sia portata a 64 miliardi di euro rispetto ai 53,4 miliardi inizialmente previsti. L'articolo 3 modifica i commi da 2 a 5 dell'articolo 11 della legge di bilancio per il 2016, relativo allo stato di previsione del Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e la consistenza organica degli allievi delle scuole militari. Il comma 1 dell'articolo 4 introduce il comma 35-*bis* all'articolo 17 della legge di bilancio per il 2016, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016. Tale fondo viene dotato di un miliardo di euro; le risorse non utilizzate nel 2016 potranno essere utilizzate, in conto residui, nell'esercizio successivo. Il comma 2 aumenta la dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 25 milioni di euro a 955.069.060 di euro per l'anno 2016. L'incremento si giustifica in considerazione del fatto che l'anno finanziario presenta ancora alcuni mesi cruciali prima della sua conclusione, e quindi il Governo ha scelto di adottare una linea di estrema prudenza, anche in considerazione delle gravi emergenze che hanno colpito il Paese durante l'estate e delle spese urgenti e impreviste sorte negli esercizi precedenti prima della fine dell'anno. Questa è l'analisi tecnica sui contenuti del disegno di legge di assestamento, i quali evidenziano come la crescita sia ancora lenta, debole, rispetto alle attese. Una ricetta che possa invertire l'andamento di questi dati è stata ed è oggetto di ampio dibattito, e ne abbiamo discusso anche in Commissione. È vero che l'economia internazionale influisce negativamente su quella nazionale, ma è anche vero che il nostro Paese ha la responsabilità di non aver colto in passato momenti favorevoli per avviare un processo di crescita e che solo in questi ultimi anni si è cercato di individuare un percorso coerente tra interventi sull'economia, sul sociale, sul lavoro anche attraverso riforme strutturali che possano contribuire a questo disegno di crescita. Tuttavia - come è stato più volte osservato - i frutti e i benefici di queste politiche si coglieranno nel tempo tempo e il nostro Paese ha bisogno di una politica di bilancio in grado di anticipare gli effetti attraverso stimoli più mirati alla crescita e alla creazione di occupazione. Queste politiche debbono necessariamente essere coordinate con le riforme strutturali avviate. Quindi, la riflessione a cui tutti siamo invitati va nella direzione di come oggi, nel quadro delle politiche già avviate di lungo termine, si possano immaginare questi interventi per dare una risposta positiva più ravvicinata.

La strategia di politica economica e fiscale delineata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF sarà determinante in tal senso. Se vogliamo leggere con nitidezza le parole «crescita economica» e «riduzione del debito pubblico» sui prossimi documenti economici, dobbiamo necessariamente prevedere misure che favoriscano la crescita della della ricchezza nominale, che è il vero nodo. Tali misure sono state individuate e riguardano, in particolare, il sostegno degli investimenti pubblici (possibilmente anche di quelli privati) e dei consumi.

i dati esposti dall'Assestamento di bilancio per il 2016 e dal Rendiconto del 2015 non sono positivi e ci preoccupano molto perché siamo in presenza di un quadro di finanza pubblica in peggioramento. Le previsioni per il 2017, appena esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2016, non fanno che confermare conti pubblici peggiori di quelli preventivati; previsioni che, a loro volta, tra l'altro, durante le audizioni in Commissione, Banca Italia, Corte dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio hanno definito ottimistiche, che è un eufemismo per non dire irrealistiche e forse irrealizzabili. Sembra, quindi, essersi arenato anche quell'obiettivo di crescita che tutti auspicavamo, e questo soprattutto a causa di una spesa che continua a crescere, anziché diminuire, e di una *spending review* di cui si è persa ogni traccia. È evidente, dalle cifre contenute nei documenti al nostro esame, come risulti difficile finanziare politiche di investimento e di crescita economica di fronte a una spesa che non si è riusciti sicuramente a contenere. Eppure, senza investimenti non c'è futuro. Occorre ritornare a parlare di crescita nelle politiche nazionali e soprattutto in quelle europee, che risultano trincerate ancora dentro una visione ragionieristica e contabile, e non economica e sociale. La mancata crescita, inoltre, genera un incremento della spesa pubblica soprattutto di tipo sociale tesa a sostenere le fasce più deboli, e questo imprime una accelerazione al debito pubblico che, anziché ridursi, aumenta costantemente. Purtroppo, è il classico caso del cane che si morde la coda. A mio avviso, ci sono due settori trainanti della nostra economia che meriterebbero più attenzione e sui quali si dovrebbe puntare. Il primo è l'agroalimentare, settore che cresce molto di più rispetto al PIL nazionale, e l'altro settore è il turismo che in Italia è ancora troppo legato alla stagione estiva mentre andrebbe valorizzato tutto l'anno. Un altro elemento che emerge dai documenti al nostro esame è una politica economica fatta in *deficit* con valori significativi e da cui è difficile rientrare. L'ammontare complessivo del debito è cresciuto in maniera importante, toccando nuovi *record* negativi, ed è inutile che vi dica che questo rappresenta una vera e propria ipoteca sulle nuove generazioni. Questo dovrebbe consigliare al Governo di evitare una nuova manovra in *deficit*. Al contrario, dalla Nota di aggiornamento al DEF, si annuncia una manovra con un *deficit* ancora importante, al 2,4 per cento del Pil e quindi non lontano da quello del 2016, che era al Ma emerge sopratutto che il Governo ha mancato completamente gli obiettivi di riduzione della spesa che è cresciuta in termini reali sia nel Rendiconto che nell'Assestamento. La conseguenza di queste politiche è che siamo in presenza di un elevato fabbisogno e di un dato negativo rispetto al risparmio pubblico, a conferma della crescita sopratutto delle spese correnti. Soprattutto, si è registrata una sensibile crescita della spesa per beni e consumi intermedi, cioè quella spesa la cui opacità lascia margini alla mediazione della politica. In presenza di questi dati, che è sinceramente difficile giudicare come positivi, ma anche in presenza di una clausola di salvaguardia sull'IVA per 15 miliardi di euro nel 2017 e di anticipazioni su un allentamento delle regole pensionistiche, ci viene una domanda: dove si andranno a prendere tutti questi soldi? La Nota è quindi, non a caso, ancora vaga sui contenuti della manovra di bilancio per il prossimo anno. Il risultato più evidente è che si sono sfilacciate quelle politiche di rigore sui conti pubblici, che avrebbero, tra l'altro, evocato i minori oneri pagati sul debito pubblico, dovuto alle politiche monetarie espansive a livello europeo. Aumenta il ricorso al Fondo per le esigenze indifferibili, senza però avere una chiara quantificazione delle diverse destinazioni delle risorse in esso appostate. La mancanza di politiche di sviluppo è proprio l'altro dato evidente con cui bisogna fare i conti. Ci sembra allora che tutti gli indicatori non depongano a favore, anzi rischino di compromettere la tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo, ma anche nel medio periodo, qualora mutassero le ancora favorevoli condizioni internazionali. Tra l'altro gli indicatori - come dicevo pocanzi - si rapportano a un PIL che registra una continua revisione al ribasso, anche secondo gli ultimi dati relativi al 2016. E di fronte a questo quadro a dir poco problematico non si riescono a leggere i contorni della manovra nemmeno nella Nota di aggiornamento al DEF, che dovrebbe, al contrario, servire proprio ad anticiparne i contenuti; una manovra che - secondo quanto ci preavvisano le indicazioni dei due documenti al nostro esame - non può che proseguire con un nuovo allentamento delle politiche volte al miglioramento dei conti pubblici. Non siamo i soli a paventare uno scenario poco roseo per il futuro del Paese. Purtroppo anche gli indicatori statistici, che misurano la fiducia di imprese e consumatori ci confermano che le difficoltà e la crisi sono tutt'altro che superate. Sono di ieri i dati dell'ISTAT sull'aumento della propensione al risparmio delle famiglie che, nonostante abbiano a disposizione un reddito maggiore per effetto dell'aumento del potere d'acquisto, preferiscono accantonare il loro denaro, piuttosto che spenderlo in acquisti o investimenti. Questo è il segnale tipico della paura e spetta a voi, signori del Governo, far ritornare fiducia nelle famiglie e nelle imprese. E lo si può fare se avrete verso la pubblica amministrazione, verso la gigantesca macchina dello Stato, lo stesso atteggiamento del buon padre di famiglia e soprattutto dell'imprenditore diligente.

misure di spesa pubblica, ma anche di stimolo alla crescita, consentendo agli imprenditori onesti e solidi di poter agevolmente investire nelle loro aziende e rendere le loro imprese più competitive. Confidiamo che fra pochi giorni, quando leggeremo la legge di stabilità, troveremo quelle misure che famiglie e imprese si aspettano, per poter guardare con fiducia al futuro e a un orizzonte temporale più lungo.

il Rendiconto e l'Assestamento del bilancio dello Stato, vanno inseriti nella strategia di preparazione economica pluriennale che il Governo si è dato dal momento del suo insediamento. I principali obiettivi di questa strategia sono il rilancio della crescita, dell'occupazione e degli investimenti pubblici e privati, che nel loro insieme stanno dando i primi evidenti risultati, com'è stato evidenziato anche dalla Nota di aggiornamento al DEF dello scorso aprile, il cui esame è stato appena avviato dalla Commissione bilancio. Al nostro esame abbiamo due documenti: un Rendiconto che oggettivamente rispetta le previsioni e un Assestamento che, invece, sconta il rallentamento della crescita del Paese all'interno di un più ampio rallentamento della crescita europea. Dal 2014, dopo diversi anni di contrazione della crescita, l'economia italiana è tornata a crescere e, con essa, è tornata a crescere l'occupazione. Questo percorso, tuttavia, ha subito un rallentamento nell'ultimo trimestre, sulle cui cause cui cause va aperta una riflessione che ragioni sul perché il Paese cresce di meno rispetto agli altri Paesi europei e sul perché l'Europa cresce di meno rispetto alle altre economie mondiali. Certamente ci sono cause evidenti: ci sono un peggioramento del quadro internazionale; il rallentamento delle economie emergenti; una debolezza protratta dell'eurozona, che è stata anche aggredita dalla crisi legata alla scelta della Gran Bretagna; l'accresciuta volatilità dei mercati internazionali e, non da ultimo, tutte le tutte le questioni geopolitiche gravi che stanno in qualche modo colpendo tutta l'area del Mediterraneo e che si riverberano sull'Europa. Ma questo non basta per comprendere e ragionare sino in fondo sulla tenuta del nostro Paese. Ovviamente gli elementi e gli effetti di queste valutazioni si riflettono sui dati contenuti nel disegno di legge n. 2521 (Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015), rispetto al quale penso sia opportuno - come ho detto in premessa sottolineare l'andamento positivo della gestione di competenza, che ha fatto registrare, rispetto alle previsioni, un miglioramento dei saldi, che si concretizza anche rispetto ai risultati raggiunti nel 2014. Grazie al buon andamento delle entrate finali, il saldo netto da finanziare nel 2015 presenta un miglioramento di 11 miliardi rispetto a quello del 2014 e anche il valore del risparmio pubblico presenta un andamento migliore rispetto alle previsioni, anche se naturalmente negativo (ed è giusto sottolinearlo). che questo andamento è riconducibile nettamente a un'attenzione, a un tentativo e a un'impostazione di politica fiscale che ha avuto in questi anni più anni più recenti un carattere espansivo. Sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato che abbiamo registrato nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del limite che il Parlamento ha stabilito con la legge di stabilità 2015, anche perché sono state positive le entrate finali rispetto al 2014 (specie quelle tributarie); andamento riconducibile anche agli interventi che sono stati fatti dal Parlamento in materia di semplificazione fiscale, a partire dalle scelte relative alla gestione della dichiarazione dei redditi precompilata (solo per fare un esempio). Per quanto concerne invece le spese, c'è stato un incremento di quelle correnti, come è stato anche sottolineato. Tuttavia, vorrei capire una cosa: se non si fa un incremento delle spese correnti per interventi a sostegno della crescita e della promozione dell'equità, che cos'altro si deve fare per sostenere la ripresa? Ora, rispetto alle spese, che - come dicevo - sono aumentate, il dato apparentemente negativo di riduzione delle spese in conto capitale è invece riconducibile certamente al buon esito del processo di pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione, che, sin dall'inizio di questa legislatura, era stato tra le priorità del nostro del nostro lavoro e della maggioranza di Governo. Questa è una scelta netta che ha fatto il Parlamento - e che il Governo ha realizzato - che aveva determinato nel biennio precedente un'immissione di liquidità nel sistema economico del Paese assolutamente straordinaria. Nel complesso, quindi, una nota da sottolineare rispetto ai dati del Rendiconto è certamente il fatto che, nella costruzione dei dati contabili e nella formulazione delle previsioni da parte del Governo,

confermata allo 0,8 per cento, così com'è stato garantito e pienamente centrato l'obiettivo del rapporto *deficit-*PIL, che certo non è il più efficiente in assoluto, ma è quello che era stato previsto del 2,6 per cento. Allo stesso modo era stata prevista una stabilizzazione del rapporto debito-PIL che è stata

endogeni, quanto per fattori che si sono sviluppati quest'anno e che hanno a che fare con il contesto europeo e internazionale che registra evidentemente un rallentamento globale dell'economia mondiale, i cui effetti, su un'economia come la nostra che è più fragile di altre anche in Europa, si stavano evidenziando già da tempo. Qui va sicuramente approfondita la riflessione sul che fare. La minaccia del terrorismo, la crisi delle migrazioni e la Brexit hanno avuto influenza sulla ripresa in Europa e quindi hanno influenzato negativamente anche la crescita nel nostro Paese. Sono fenomeni che hanno una portata

Troppo debole, troppo prudente e troppo timorosa è stata la strada che sino a questo momento l'Europa ha portato avanti. Lo dimostrano anche l'inefficacia la portata minima del Piano Juncker, nonostante l'Italia sia il secondo tra i Paesi europei che stanno cercando di investire su tale piano, con 13 progetti sinora approvati e inseriti. Ciò dimostra che l'Europa non sta facendo sufficientemente per proteggere la propria crescita

dire, se si guarda più avanti nel tempo, ai prossimi venti anni, che il rischio che l'economia europea diventi assolutamente marginale rispetto ad altre economie emergenti è una realtà alla quale guardare con grave preoccupazione e rispetto alla quale un solo Paese, per di più fragile come il nostro, non può dare certamente la sterzata che sarebbe necessaria. Può invece contribuire a una direzione di marcia il tentativo che il Parlamento e il Governo stanno facendo con la Commissione europea, finalizzato a consolidare a quel livello un'azione di sostegno alla crescita e all'occupazione attraverso un'incentivazione delle politiche di investimenti e di riforme che cambino in modo strutturale le potenzialità e il lavoro che l'Europa sta facendo in quella direzione. Sono sufficienti? No, perché l'Europa non sta ancora andando nella direzione che serve, ma in ogni caso quella è l'unica direzione nella quale Parlamento e il Governo, con il sostegno di tutto il Parlamento nel suo insieme, devono procedere. Nonostante questa economia e questo quadro economico ancora deboli, l'indebitamento del Paese si è mantenuto sotto il limite del 3 per cento e in termini strutturali siamo ormai molto vicini al pareggio di bilancio. Non voglio citare ora tutto il resto dei temi che riguardano specificamente l'Assestamento. Vado invece ad alcuni dati conclusivi e di sintesi che ritengo siano importanti. Penso sia importante segnalare che il rallentamento della crescita nel 2016 e, come si vede già dalla Nota di aggiornamento del DEF, nel 2017, colpisce molte delle economie europee e richiede una riflessione che certamente dobbiamo fare in sede di discussione della legge di stabilità e della prossima legge di bilancio, inserendo misure a favore della crescita e rivolte al superamento delle disuguaglianze che colpiscono in maniera più evidente ed espone alla crisi i soggetti più deboli e coloro che hanno minori risorse materiali e immateriali. Ma è il sistema Paese nell'insieme che richiede un'innovazione e una capacità di investire maggiormente su se stesso e sulle proprie risorse. In questi anni si è lavorato si è lavorato molto nella direzione della riduzione delle imposte in maniera diffusa, per aumentare la disponibilità di risorse per le famiglie e per le persone, dobbiamo fare in modo che questa disponibilità di risorse si tramuti, attraverso un'iniezione di fiducia, in consumi e investimenti. Non condivido alcune

se nel 2016 stiamo registrando alcuni scostamenti, questi sono legati a fattori sicuramente esterni. Così come c'è stata la riduzione della spesa primaria (siamo a livello di pareggio di bilancio strutturale), ma non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, pretendendo di avere più investimenti e nello stesso tempo di investire meno risorse.

signor vice ministro Morando, colleghi, l'esame del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 e della Nota di aggiornamento

di tre Governi che negli ultimi cinque anni si sono succeduti alla guida del Paese: i Governi Monti, Letta e Renzi. Cinque anni equivalgono a una legislatura piena credo che i risultati prodotti siano sotto gli occhi di tutti e siano fallimentari. Le politiche economiche di questi Governi hanno portato una larga fetta degli italiani alla disperazione. I parametri economici più significativi, quelli che possono consentire una puntuale valutazione dell'azione del Governo, purtroppo sono tragici. Il debito pubblico, tra il novembre 2011 e il luglio 2016, data dell'ultima certificazione della Banca d'Italia, è cresciuto di 350 miliardi di euro.

i debiti accumulati dalla pubblica amministrazione nei confronti delle aziende: se lo Stato avesse pagato le aziende per circa 70 miliardi, il debito pubblico sarebbe emerso in maniera ancora più rilevante.

spera - ma nella sostanza chiudono le aziende, abbiamo -25 miliardi di produzione industriale e -30 miliardi di investimenti fissi lordi. Questi Governi, che dovevano mettere i conti in ordine, in realtà, stanno mettendo a soqquadro il Paese. Il pareggio di bilancio, che il Governo Monti aveva fissato al 2013,

dal consuntivo e arriverà al 132,8 per cento alla fine del 2016. Ma, tranquilli, non vi preoccupate: l'anno prossimo inizierà a scendere! la disoccupazione, ad agosto la stima degli occupati registra un lieve incremento, passando, a luglio, a +0,1 con 13.000 occupati in più, dopo il calo registrato nel mese precedente, dello 0,3 per cento con 40.000 occupati in meno. Il tasso di disoccupazione è pari all'11,4

In dieci anni le famiglie italiane che vivono in povertà assoluta sono quasi raddoppiate, passando da 819.000 del 2005 a 1,5 milioni nel 2015. Gli individui in grave difficoltà sono addirittura aumentati del 140 per cento, passando da 1,9 milioni a 4,6 milioni. Al 31 dicembre 2015 la popolazione con cittadinanza italiana è scesa di 179.000 unità. Le nascite sono state 488.000 ed è il minimo storico dall'Unità d'Italia a oggi: per il quinto anno consecutivo

è uno sforzo che il Paese deve fare, non può far fuggire all'estero tutti i cervelli formati dalle università italiane! Il Governo deve assolutamente far ripartire la crescita, e la crescita non riparte

e facilitando l'accesso al credito, che ormai è completamente chiuso perché le banche sono tutte in difficoltà. Dobbiamo aiutare le aziende che hanno voglia di fare ricerca e innovazione, sviluppando e acquistando

Di fronte a questa tragica situazione, continuate a prendere in giro gli italiani. Questo consuntivo dimostra che le vostre previsioni sono sistematicamente, dieci volte su dieci, prive di fondamento. Alla prova dei fatti si dimostrano completamente errate: previsioni che vengono fatte per illudere, ma, di illusione in illusione, il Paese precipita nel baratro, perché continuando a fare previsioni sballate non facciamo altro che aumentare il debito pubblico, perché l'anno successivo vi è sempre un*surplus* di debito pubblico. Non siete riusciti neanche a sfruttare una congiuntura internazionale favorevole, quale è stata quella del costo del denaro pari a zero,

la riduzione del costo del denaro non durerà in eterno; il petrolio ha già cominciato a salire e le previsioni del prezzo del petrolio contenute nella Nota di aggiornamento al DEF sono completamente sballate, sono già fuori misura. Il commercio internazionale, che può sostenere la nostra economia, dovrà fare i conti con una crisi che lo sta riducendo. Avviandomi alla

a dare un'informazione adeguata, perché non possiamo ancora operare

ponga fine, dopo cinque anni, a una stagione fatta di promesse non mantenute e di favole, perché il Paese ha bisogno di un Governo che dica con chiarezza agli italiani come stanno le cose. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà. Signor Presidente, mi ha appassionato l'intervento del collega Ceroni, perché ha centrato l'obiettivo della discussione di oggi. Leggere un bilancio è un po' un valzer di numeri. Il bilancio è la conseguenza di scelte politiche, valutazioni e previsioni, per lo più;

che abbiamo dovuto fare ben sette revisioni e sette sanatorie per sanare blocchi di persone che risultavano non comprese (mi riferisco ai famosi esodati) nel precedente provvedimento.

può preventivare eventi sismici come quelli avvenuti nel corso dell'anno o, per esempio, le alluvioni degli anni scorsi. Del resto, non possiamo non ricordare che tutte le Regioni del Nord,

credere al Governo quando afferma che siamo in ripresa, che c'è crescita, se il dato della produzione industriale è stagnante.

se lo vogliamo fare adesso, ahimè, sappiamo che facciamo solo facile e facilissima propaganda.

non possiamo parlare di lavoro agile, perché esso non è possibile. C'è un rapporto tanto stretto tra datore di lavoro

alle persone che tutto va bene e che le tasse diminuiscono, perché ogni singolo cittadino fa i propri conti e vede che è sempre più impoverito!

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, ancora una volta ci troviamo a esaminare documenti di bilancio

lo stato di difficoltà in cui il Paese si trova e l'incapacità del Governo nel porvi rimedio. Se dovessimo raffrontarli ognuno al suo contesto, ossia il Rendiconto, che prende le mosse dal

dei documenti. Infatti, abbiamo sempre previsioni in eccesso e abbiamo sempre una legge di stabilità che privilegia l'aumento della spesa pubblica e molto spesso, come accade da due anni a questa parte, la privilegia nel senso di accattivarsi la benevolenza Oggi siamo in scadenza della data referendaria e, quindi, ci attendiamo, ancora una volta, una legge di stabilità ricolma di proposte accattivanti. Magari poi, nel combinato disposto delle date, qualcuno si renderà conto che le proposte accattivanti possono anche svanire dinanzi a un risultato negativo dello stesso *referendum*. Ci troviamo di fronte a questa sequenza di documenti che purtroppo evidenza lo stato di assoluta difficoltà della nostra economia, che però in larga parte non è dovuto a fattori esterni, come i colleghi della maggioranza più volte si sono premurati di evidenziare e che sicuramente ci sono. Per la verità, in questi ultimi anni i fattori esterni sono stati più favorevoli a una spinta dell'economia italiana: dalla diminuzione del prezzo del petrolio, al cambio con il dollaro, ai tassi internazionali, a tutta una serie di contingenze che in altri contesti e, soprattutto, con un'altra guida governativa avrebbero potuto consentire risultati positivi.

di alcuni indicatori e del fatto che, ogni tanto, anche gli istituti di rilevazione, dopo aver espresso dati negativi, si affrettano, evidentemente adeguatamente sollecitati, a cercare di dire qualcosa che possa essere migliorativa rispetto al passato. La verità è che, se aumenta

il Governo preannuncia, sempre nell'ambito di quella *captatio benevolentiae* dell'elettorato che ritiene assolutamente indispensabile da perseguire in questa fase, addirittura un condono fiscale fiscale e la possibilità di una rottamazione dei ruoli. Può darsi che abbia intercettato il desiderio di una parte del nostro elettorato a essere

che un provvedimento di questo tipo sicuramente sarebbe utile alle casse dello Stato e a un rasserenamento dei rapporti tra cittadino

a scopi ben diversi dal risanare i conti dello Stato e promuovere l'aumento della produttività del Paese. L'aumento della produttività non solo è azzerato, ma direi che è addirittura crollato e in maniera evidente. Abbiamo visto i dati sugli ordinativi industriali negli ultimi mesi e tutta una serie di dati

per non parlare degli Stati emergenti nel panorama economico mondiale. Siamo sempre fanalino di coda e lo siamo ancora di più, purtroppo, in questo momento. Discuteremo tra poco il Documento di economia e finanza e anche in naturalmente, ci scontreremo su previsioni che noi riteniamo assolutamente fuori dalla realtà, come le ritengono anche gli osservatori terzi che abbiamo ascoltato: la Banca d'Italia, la Corte dei conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

due anni fa ad un clamoroso scippo, perpetrato nei confronti del Mezzogiorno, di oltre 4,5 miliardi di risorse destinati ad investimenti e utilizzati per la decontribuzione delle nuove assunzioni, inizia a segnare il passo, perché quest'anno si è dovuta ridurre al 40 per cento, e che tra due anni ci regalerà una bolla occupazionale di grandissime proporzioni. Infatti, quelle decontribuzioni non sono state legate

"furbette" nell'utilizzare gli incentivi che i Governi ammanniscono, utilizzeranno per tre anni la decontribuzione e, non avendo alcun obbligo e non avendo ricavato alcun aumento della produttività, perché questo ci dicono i dati,

la ringrazio per avermelo consentito, perché credo che questa riflessione sull'Assestamento di bilancio non possa prescindere dalla realtà e da quello che accade intorno a noi. È vero che stiamo

cosa accadrà ai fini del bilancio dello Stato - e questo è il nesso del mio intervento - rispetto a ciò che si sta verificando, appunto, nel mondo bancario. Ieri è stato lanciato un grido d'allarme da un autorevolissimo giornalista italiano, Ferruccio De Bortoli, il quale ha scritto un articolo che è un'inchiesta più che un editoriale, sul «Corriere della Sera» cui oggi ha risposto, per certi versi, il Ministro dell'economia

con interferenze pubbliche. Quindi noi, al di là del minuetto sull'Assestamento, sul bilancio e su quello che discutiamo, dobbiamo andare alla sostanza dei problemi perché - come ha scritto ieri De

termine che francamente non riesco ad associare al Ministro dell'economia, soprattutto ad una figura così austera e severa come Padoan - e da facilitatore (di non si sa che cosa) sarebbe intervenuto per comunicare che doveva cambiare l'amministratore del Monte dei Paschi di Siena. Il Tesoro ha solo il quattro per cento di questa banca quotata in borsa, tanto è vero che questo intervento così improprio di chi deve poi gestire i conti, l'assestamento, il rigore finanziario - a cui ci si richiama tutti i giorni

Dopodiché, però, molti di questi problemi si sono verificati anche quando alcune operazioni relative al Monte dei Paschi di Siena

ne verrebbe fuori un miliardo. Siccome vedo che ogni tanto facciamo annunci del tipo: un miliardo per le pensioni, un miliardo per quello, rinnoviamo i contratti, assestiamo il bilancio, non è una vicenda estranea. Pertanto, dico

siamo contrari all'assestamento della manovra. Non possiamo contestare che due più due fa quattro: sarà tutto corretto nella colonna dei numeri. Il problema è cosa succede di queste cifre. C'è una realtà occulta di debiti, di esposizioni, che può essere un costo? Quindi, stiamo approvando l'assestamento di un bilancio che potrebbe essere dissestato da vicende che riguardano il bilancio di questi anni.

tutte queste cifre dove stanno? Quanto costa? Che cosa succederà? Stiamo approvando un Assestamento assestante o un Assestamento dissestante, dissestato e con omissioni? Questo è ciò che mi chiedo. Tutto ciò che viene denunciato

Signor Presidente, le entrate e le spese individuate nel Rendiconto, nonché le modifiche proposte in assestamento, sono il risultato delle politiche economiche definite nella legge di stabilità e in generale nel DEF. Evitando di mettere in rilievo gli aspetti legati ai numeri, che sono già stati citati ampiamente, per noi il complesso dei dati esposti è assolutamente insoddisfacente rispetto alla condizione reale del Paese, alla condizione dei conti pubblici e, più in generale, alle sfide che ci attendono. Critichiamo la scarsa accuratezza delle previsioni di bilancio, che ha portato a sostanziali modifiche in sede di assestamento e l'eccessivo ottimismo, che ha fatto da cornice alla costruzione di bilancio per l'anno in corso. Le vostre politiche economiche, fiscali e di bilancio sono frutto di un perseguimento di obiettivi basati su sterili indici nominali quali il PIL. Questo indice, come tutti gli indici matematici, è sterile, perché non fa alcuna differenza tra merci e beni. Ed è evidente che la differenza esiste, eccome se esiste. Le merci sono «oggetti o servizi che si acquistano scambiandoli con denaro», mentre i beni sono «oggetti o servizi che rispondono a un bisogno». Ci siamo spesi per far introdurre gli indici di benessere equo e sostenibile, ovvero indici che contengono variabili reali tra cui la disoccupazione, la qualità della vita, l'inquinamento, fra gli obiettivi programmatici da perseguire, ma la maggioranza ha bocciato questa possibilità. Ci siamo battuti perché investimenti produttivi fossero fatti nel nostro Paese, ma, per l'urgenza di contenimento dei conti pubblici e il vostro rigoroso rispetto delle regole europee, sono state sacrificate politiche pubbliche vitali come gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche che mirano a quel benessere sociale di cui ha bisogno la collettività. Mi verrebbe da dire che, però, sulle grandi opere questo Governo ha grandi progetti! Ci siamo spesi e ci spendiamo per istituire un reddito di cittadinanza, il modello sociale europeo che l'Italia ignora. Ci appare assolutamente incomprensibile che non si ponga alcuna attenzione ai sussidi di disoccupazione europei, nonostante l'Europa ci raccomandi dal lontano 1992 di introdurre un reddito di cittadinanza (e ciò non succede neanche con la crisi). In tutti i Paesi dell'Europa questo è realtà. Non in Italia e in Grecia. D'altro canto, il Governo insiste nel sostenere che l'origine della gracilità e della debolezza della ripresa italiana è sicuramente imputabile a fattori strutturali che riguardano il nostro Paese. Sempre il Governo afferma che abbiamo un cattivo funzionamento di quelle che gli economisti chiamano le istituzioni economiche fondamentali, riferendosi al processo di formazione del capitale umano, alla giustizia, ai mercati regolati in maniera insoddisfacente e, soprattutto, all'instabilità politica, indicata come la principale colpevole dei fattori fondamentali di depressione delle nostre capacità competitive a paragone con gli altri Paesi. Dato che un Governo non dovrebbe mai e poi mai promuovere riforme costituzionali, da parte nostra invece riteniamo che la qualità delle istituzioni conti molto, più delle tanto invocate riforme. Peccato che la qualità istituzionale italiana sia lontana anni luce non solo da quella dei virtuosi Paesi del Nord Europa, ma anche dalla media dell'area euro. E infatti le economie dei Paesi in cui sono più scarsi sono più scarsi l'efficacia dell'azione del Governo, la capacità di varare e mettere in pratica leggi per promuovere lo sviluppo economico, il rispetto del principio di legalità e il controllo sulla corruzione tendono a ristagnare e, senza istituzioni forti, vincono le *lobby*. Quindi, mettere mano alle riforme non basta per rilanciare la tanto agognata crescita. Prima di mettere mano alle regole Prima di mettere mano alle regole sui contratti di lavoro, di liberalizzare i mercati e di modificare la Costituzione, occorre riformare l'ossatura del sistema, partendo dalla base: rispetto delle leggi e repressione dei reati, a partire dalla corruzione. In definitiva, abbiamo due diverse prospettive di vedere i problemi, con un ordine di priorità totalmente differente; ma il vero problema di fondo è la necessità di cambiare quel paradigma culturale che ci ha portato al dissesto, sociale e morale prima ancora che economico. L'economia non è una scienza esatta, ma è stata assunta come verità incontrovertibile e come motore di sviluppo unico del benessere sociale. Il fallimento di questo modello ci è davanti agli occhi con tutta la sua gravità. Un modello culturale che avrebbe dovuto assicurare un benessere diffuso ha generato tutto il contrario: una concentrazione di ricchezza senza precedenti nella storia, una drammatica povertà a tutti i livelli, un degrado morale e spirituale, un livello di individualismo e di conflittualità permanente, che ha disgregato il sistema sociale, a partire della famiglia, e lasciato i giovani senza prospettive future, sia in termini di valori che economiche. La crisi dipende da uomini e non da eventi naturali ed imprevedibili. Che responsabilità hanno questi uomini? Concludo. Gli economisti hanno costruito un modello basato sulla crescita infinita; ma è chiaro che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito. Quindi è naturale avvicinarsi all'idea di decrescita e cercare di trovare nuove soluzioni alla realtà che ci circonda. E la decrescita non è la crescita negativa; quest'ultima è quella che stiamo vivendo oggi e che produce disoccupazione, meno finanziamenti per la cultura, per la salute e per l'ambiente. La decrescita è uno slogan provocatorio, che serve a spiegare la necessità di rompere definitivamente con gli schemi sui quali questa società si fonda, per poter uscire dalla fede del mercato, rimettendo al centro la persona, e dalla religione dello sviluppo a tutti i costi, creando un futuro sostenibile.

In questi giorni la General Electric ha informato le istituzioni e i lavoratori della volontà di chiudere lo stabilimento di Sesto San Giovanni. È chiaro che la chiusura non avviene per una crisi industriale, ma per un processo di ristrutturazione che mira a chiudere uno stabilimento e a riutilizzare altrove i brevetti e il *know how* che in quello stabilimento sono stati costruiti. Tenendo conto che la General Electric ha ricevuto dallo Stato diversi incentivi per investire in Italia, trovo grave che in questi giorni, dopo quell'annuncio e dopo che il Governo ha aperto un tavolo di trattativa presso il Ministero dello sviluppo economico, la stessa abbia abbandonato quel tavolo, dimostrandosi indisponibile a qualunque tipo di trattativa; tavolo, quello aperto dal Governo, sostenuto con il contributo dei sindaci del territorio e dei sindacati. Il tavolo era stato aperto al Ministero dello sviluppo economico proprio perché l'obiettivo non era quello semplicemente di

Governo la richiesta di insistere e costringere General Electric a ritornare al tavolo per salvaguardare gli oltre 200 posti di lavoro di quello stabilimento, ma soprattutto per salvaguardare uno stabilimento importante per la città di Sesto San Giovanni e per il territorio del Nord di Milano. Sappiamo che il Governo si è impegnato molto in questi anni per salvaguardare il nostro apparato industriale e produttivo e credo che da questo punto di vista sia utile e importante continuare in questa direzione, tenendo aperto quel tavolo. ammissibile che un soggetto importante come General Electric, che ha ricevuto significativi incentivi per investire in Italia, possa fare scelte come quella di chiudere una fabbrica e portare via *know how* e brevetti, ma soprattutto non è tollerabile l'atteggiamento di chiusura che mostra General Electric. grave che si siano alzati dal tavolo, ma ancor più grave è l'aver impedito al sindaco di Sesto San Giovanni di portare ai lavoratori in agitazione la solidarietà della città.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Nella notte fra il 28 e il 29 settembre, a Valenza, la mia città, in Provincia di Alessandria, Rita Giuseppa Lercara, sessantasette anni, è stata uccisa a coltellate. Per l'omicidio è stato arrestato il marito. è la quindicesima donna che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno scorso. La conoscevo, anche se negli ultimi tempi non mi era più capitato di incontrarla, anche perché Valenza è una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Non solo: con lei e il suo primo marito, dal quale era rimasta vedova ormai molti anni fa, ho condiviso anche, nel corso degli anni Novanta, un tratto di militanza politica comune. Rita Lercara aveva trascorso la sua vita lavorativa nell'ambito della pubblica amministrazione locale, dedicandosi alla cura degli anziani ospiti della casa di riposo: un'attività svolta con dedizione e affetto nei confronti dei suoi assistiti.

E ancora, è rimasta vittima di stupro a Colle Oppio, proprio in questi giorni, una giovane donna australiana; una violenza subita che, per il luogo in cui è avvenuta, sta in quel sul totale dei casi di stupro di cui le donne sono vittime, che maggiormente arrivano all'attenzione dell'opinione pubblica perché avvengono in spazi pubblici e aperti, ma che non devono farci dimenticare l'enorme casistica di stupri che le donne subiscono in ambito domestico. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Nonostante, anche nel caso di Rita Giuseppa Lercara, i giornali parlino di un possibile *raptus* di follia, il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. E mi si lasci dire che è sconcertante constatare come in questo contesto, già così grave, da alcune trasmissioni anche di grande *audience* come il «Grande Fratello» su Canale 5, per responsabilità di taluni irresponsabili, arrivino anche messaggi che in qualche modo legittimano il comportamento di femminicidio. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne, e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Riproponiamo perciò con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra con delega per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 199 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata attuazione del piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi

infatti accertata dagli organi sanitari competenti, ed è purtroppo ancora in corso nella Regione Veneto, un'epidemia di febbre catarrale degli ovini, una malattia infettiva.

spaventa per i riflessi sia sulle transazioni commerciali dovute al blocco della movimentazione degli animali, disposto dalle autorità sanitarie competenti, sia ovviamente per i danni diretti alle greggi. Quindi si tratta di un'economia che subisce veramente un grande danno.

l'orientamento a coprire solo i costi per l'intervento vaccinale sui capi ovini e caprini, con la mancata estensione ai capi bovini, pongono in seria difficoltà gli allevatori.

oppure se sia stato il Ministero della salute a dare queste indicazioni. Credo sia fondamentale e importantissimo capire la filiera decisionale e perché si sia deciso di intervenire con i vaccini su alcuni capi e non su altri. Come dicevo, il virus continua a diffondersi creando non poche perdite e difficoltà ai nostri allevatori. E se è vero che il virus non colpisce le persone, che quindi si sentono al sicuro,

Signor Presidente, vorrei sottolineare e portarvi a conoscenza di un ennesimo episodio di scempio ambientale e dei posti di lavoro che, viceversa, potremmo creare con le bonifiche e con la produzione *green*.

tra l'altro, hanno trovato anche traversine ferroviarie. Le banali traversine ferroviarie che però tanto banali non sono, perché contengono olio di creosoto, una miscela di composti chimici derivati dalla distillazione del catrame di carbone, con cui le traversine venivano impregnate per aumentarne le caratteristiche di durabilità.

clinici ed epidemiologici, che hanno stabilito definitivamente la cancerogenicità del benzopirene contenuto. In poche parole, il creosoto è estremamente tossico: molti suoi componenti sono bioaccumulabili e la degradazione di questi elementi è molto lenta

Tali considerazioni non sono certamente mie, ma ribadite dalla Commissione europea che lo ha dichiarato in un apposito comunicato. Ovviamente noi condanniamo totalmente e incondizionatamente gli autori di questo smaltimento illecito e, viceversa, lodiamo l'operato della Guardia di finanza in questo tipo di interventi.

Guardando al futuro, invece, questo dovrebbe esortarci per l'ennesima volta a produrre misure di politica industriale - che invece mancano - volte ad agevolare la creazione di altrettante decine di migliaia di posti di lavoro per passare dalla pericolosissima, mortale, petrolchimica alla chimica verde, di cui proprio sabato scorso abbiamo avuto un picco positivo positivo con l'inaugurazione di una bioraffineria. Peccato che questa sia un caso eccezionale e non la norma. Come Movimento 5 Stelle, se fossimo al Governo, invertiremmo questa situazione e l'apertura di fabbriche pulite, operanti con la modalità dell'economia circolare, di cui troppi si riempiono la bocca, diventerebbe la regola e non l'eccezione. Il Governo, invece, cosa fa? Annuncia il *green* *act* e poi, miseramente, tace.

Grazie